In data 10 marzo 2023 è stato presentato il seguente disegno di legge: dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell’interno, dal Ministro della giustizia, dal Ministro degli affari esteri e della coopera- zione internazionale, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Mi- nistro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste «Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare» (591). Comunico che nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna è pubblicato l’elenco dei senatori e dei deputati chiamati a far parte della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

che il Governo proclami innanzitutto lo stato di emergenza. Un’altra parte dell’Umbria, quella dell’alta Valle del Tevere, in particolare il Comune di Umbertide, nelle frazioni di Pierantonio e Pian d’Assino, e anche in parte la zona di Perugia, con le frazioni di Sant’Orfeto e Cenerente, sono state colpite da un evento sismico nei giorni scorsi. Sono circa 500 gli sfollati e quelle realtà così popolose, produttive, molto legate anche alla mobilità - si tratta di aree che insistono lungo la E45

le modalità per dare risposte più rapide. Qualcuno parla di un provvedimento ad hoc - per il quale saremmo disponibili anche noi come Partito Democratico - di allargamento del cratere anche a quelle tre realtà.

infine la nostra solidarietà sincera a quei cittadini, agli amministratori locali, ai tecnici, alla Protezione civile, alla Croce Rossa, a tutti coloro che in queste ore sono sul campo, chiediamo davvero che il Governo faccia prima possibile a dare segnali di fiducia a quelle popolazioni.